che ieri è scomparso a Napoli l'onorevole Giovanni Roberti, parlamentare per molte legislature. Egli apparteneva a quella generazione nitidamente missina e corporativa che aveva addirittura preceduto i parlamentari della generazione di mio padre, di cui, con diversi sentimenti etico-civili, era stato collega, oltre che alla Camera dei deputati, alla facoltà di scienze politiche. Egli era un benemerito degli studi di diritto del lavoro, ovviamente della tradizione fascista fascista e corporativa anteriore a quella che fu la generazione dei Giugni e dei Mancini, per non parlare di quella odierna giunta su posizioni liberali e liberiste. L'onorevole Roberti è stato un uomo che alla città di Napoli, oltre che alla sua parte politica, ha sempre dato dignità ed eleganza di stile. Nella sua vecchiaia non ha mai fatto mancare, nelle prese di posizione pubbliche, un sentimento civile di amore alla città, alla propria bandiera e al proprio Paese.

Carofiglio. Nel giorno in cui la Corte europea dei diritti dell'uomo dichiara inammissibile il ricorso di un Ministro del I Governo Berlusconi, condannato con sentenza definitiva per corruzione aggravata, così riconoscendo l'equità del giudizio cui egli è stato sottoposto, la maggioranza si accinge ad un ulteriore, devastante passaggio del suo cinico progetto di disarticolazione della giustizia italiana. Al dispiegarsi di questo cinico progetto assiste un pubblico esterrefatto e sgomento di avvocati, di personale giudiziario, di magistrati, di professionisti della sicurezza e soprattutto di cittadini. Mentre questa maggioranza - tristemente ridotta al rango di mera esecutrice di ordini - parla di dialogo, rifiuta con cocciuta e inquietante determinazione ogni ipotesi di miglioramento del testo in discussione, rendendo drammaticamente trasparenti le vere ragioni del suo procedere. Vi è uno scenario che si intravede alla fine di questo percorso. Questo scenario è né più né meno che lo scempio della giustizia italiana. Lasciatemelo ripetere: lo scempio della giustizia italiana. Di questo scempio vi assumete davanti al Paese tutta la responsabilità politica e morale.

...condannato con sentenza definitiva per corruzione aggravata, così riconoscendo l'equità del giudizio cui egli è stato sottoposto, la maggioranza si accinge ad un ulteriore devastante passaggio del suo cinico progetto di disarticolazione della giustizia italiana. Al dispiegarsi di questo cinico progetto assiste un pubblico esterrefatto e sgomento di avvocati, di personale giudiziario, di magistrati, di professionisti della sicurezza e, soprattutto, di cittadini. Mentre questa maggioranza - tristemente ridotta al rango di mera esecutrice di ordini - parla di dialogo, rifiuta con cocciuta e inquietante determinazione ogni ipotesi di miglioramento del testo in discussione, rendendo drammaticamente trasparenti le vere ragioni del suo procedere. Vi è uno scenario che si intravede, alla fine di questo percorso. Questo scenario è né più né meno che lo scempio della giustizia italiana. Lasciatemelo ripetere: lo scempio

riguardante la corruzione e la truffa ai danni dello Stato, proposta portata avanti non da me o dai miei colleghi, ma dall'intero Comune di Milano, compreso il sindaco Moratti. a leggere anch'io la seguente dichiarazione di voto. Nel giorno in cui la Corte europea dei diritti dell'uomo dichiara inammissibile il ricorso di un Ministro del I Governo Berlusconi, condannato con sentenza definitiva per corruzione aggravata, così riconoscendo l'equità del giudizio cui egli è stato sottoposto, la maggioranza si accinge ad un ulteriore, devastante passaggio del suo cinico progetto di disarticolazione della giustizia italiana. Al dispiegarsi di questo cinico progetto assiste un pubblico esterrefatto e sgomento di avvocati, di personale giudiziario, di magistrati, di professionisti della sicurezza e soprattutto di cittadini. Mentre questa maggioranza - tristemente ridotta al rango di mera esecutrice di ordini - parla di dialogo, rifiuta con cocciuta e inquietante determinazione ogni ipotesi di miglioramento del testo in discussione - come risulta dall'esempio citato poc'anzi rendendo drammaticamente trasparenti le vere e uniche ragioni del suo procedere. Vi è uno scenario che si intravede alla fine di questo percorso. Questo scenario è né più né meno che lo scempio della giustizia italiana. Lasciatelo ripetere anche a me: lo scempio della giustizia italiana. Di questo scempio vi assumete davanti al Paese tutta la responsabilità politica e morale.

in cui la Corte europea dei diritti dell'uomo dichiara inammissibile il ricorso di un Ministro del I Governo Berlusconi, condannato con sentenza definitiva per corruzione aggravata, così riconoscendo l'equità del giudizio cui egli è stato sottoposto. La maggioranza oggi si accinge, nonostante questo precedente significativo, ad un ulteriore, devastante passaggio del suo cinico progetto di disarticolazione della giustizia italiana. Al dispiegarsi di questo cinico progetto assiste un pubblico esterrefatto e sgomento di avvocati, di personale giudiziario, di magistrati, di professionisti della sicurezza e soprattutto di cittadini, quei cittadini a nome dei quali avete - in maniera Mentre questa maggioranza, tristemente ridotta al rango di mera esecutrice di ordini - sì, insisto parla di dialogo, rifiuta con cocciuta ed inquietante determinazione ogni ipotesi di miglioramento del testo in discussione, rendendo drammaticamente trasparenti le vere ragioni del suo procedere. Vi è quindi uno scenario che si intravede alla fine di questo percorso. Questo scenario è né più né meno che lo scempio della giustizia italiana. Lasciatemelo ripetere: è lo scempio della giustizia italiana. Di questo scempio vi assumete davanti al Paese tutta la responsabilità politica e morale.

anch'io la dichiarazione che hanno letto i miei colleghi poc'anzi. Nel giorno in cui la Corte europea dei diritti dell'uomo dichiara inammissibile il ricorso di un Ministro del I Governo Berlusconi, condannato con sentenza definitiva per corruzione aggravata, così riconoscendo l'equità del giudizio cui egli è stato sottoposto, la maggioranza si accinge ad un ulteriore, devastante passaggio del suo cinico progetto di disarticolazione della giustizia italiana. Al dispiegarsi di questo cinico progetto assiste un pubblico esterrefatto e sgomento di avvocati, di personale giudiziario, di magistrati, di professionisti della sicurezza e, soprattutto, di cittadini. Mentre questa maggioranza parla di dialogo, rifiuta con cocciuta ed inquietante determinazione ogni ipotesi di miglioramento del testo in discussione, rendendo drammaticamente trasparenti le vere ragioni del suo procedere. Vi è uno scenario che si intravede alla fine di questo percorso: questo scenario è né più né meno che lo scempio della giustizia italiana. Lo ripeto: lo scempio della giustizia italiana. Di questo scempio vi assumete davanti al Paese tutta la responsabilità politica e morale.

Signora Presidente, leggero anch'io la dichiarazione che hanno letto i miei colleghi. Signori del Governo,nel giorno in cui la Corte europea dei diritti dell'uomo dichiara inammissibile il ricorso di un Ministro del I Governo Berlusconi, condannato con sentenza definitiva per corruzione aggravata, così riconoscendo l'equità del giudizio cui è stato sottoposto, la maggioranza si accinge ad un ulteriore, devastante passaggio del suo cinico progetto di disarticolazione della giustizia italiana. Al dispiegarsi di questo cinico progetto assiste un pubblico esterrefatto e sgomento di avvocati, di personale giudiziario, di magistrati, di professionisti della sicurezza e soprattutto di cittadini. Mentre questa maggioranza - tristemente ridotta al rango di mera esecutrice di ordini - parla di dialogo, rifiuta con cocciuta e inquietante determinazione ogni ipotesi di miglioramento del testo in discussione, rendendo drammaticamente trasparenti le vere ragioni del suo procedere. disarticolazione della giustizia italiana. Vi è uno scenario che si intravede alla fine di questo percorso. Questo scenario è né più né meno che lo scempio della giustizia italiana. Lasciatemelo ripetere: lo scempio della giustizia italiana. Di questo scempio vi assumete davanti al Paese tutta la responsabilità politica e morale.

il fatto, che riteniamo gravissimo, che nel giorno in cui la Corte europea dei diritti dell'uomo dichiara inammissibile il ricorso di un Ministro del I Governo Berlusconi, condannato con sentenza definitiva per corruzione aggravata, così riconoscendo l'equità del giudizio cui egli è stato sottoposto, la maggioranza si accinge ad un ulteriore, devastante passaggio del suo cinico progetto di disarticolazione della giustizia italiana. Vi è uno scenario che si intravede alla fine di questo percorso. Questo scenario è né più né meno che lo scempio della giustizia italiana. Lasciatemelo ripetere: lo scempio della giustizia italiana. Di questo scempio vi assumete davanti al Paese tutta la responsabilità politica e morale. *(Applausi dal

così riconoscendo l'equità del giudizio cui egli è stato sottoposto, la maggioranza si accinge ad un ulteriore, devastante passaggio del suo cinico progetto di disarticolazione della giustizia italiana. Al dispiegarsi di questo cinico progetto assiste un pubblico esterrefatto e sgomento di avvocati, di personale giudiziario, di magistrati, di professionisti della sicurezza e, soprattutto, di cittadini. Mentre questa maggioranza - tristemente ridotta al rango di mera esecutrice di ordini - parla di dialogo, rifiuta con cocciuta e inquietante determinazione ogni ipotesi di miglioramento del testo in discussione, rendendo drammaticamente trasparenti le vere ragioni del suo procedere. Vi è uno scenario che si intravede, alla fine di questo percorso. Questo scenario è né più né meno che lo scempio della giustizia italiana. Lasciatemelo ripetere: lo scempio della giustizia italiana.

rifiuta con cocciuta e inquietante determinazione ogni ipotesi di miglioramento del testo in discussione, rendendo drammaticamente trasparenti le vere ragioni del suo procedere. Vi è uno scenario che si intravede alla fine di questo percorso. Questo scenario è né più né meno che lo scempio della giustizia italiana. Lasciatemelo ripetere: lo scempio della giustizia italiana. Di questo scempio vi assumete davanti al Paese tutta la responsabilità politica e morale.

Nel giorno in cui la Corte europea dei diritti dell'uomo dichiara inammissibile il ricorso di un Ministro del I Governo Berlusconi, condannato con sentenza definitiva per corruzione aggravata, così riconoscendo l'equità del giudizio cui egli è stato sottoposto, la maggioranza si accinge ad un ulteriore, devastante passaggio del suo cinico progetto di disarticolazione della giustizia italiana.

cittadini. Mentre questa maggioranza - tristemente ridotta al rango di mera esecutrice di ordini - parla di dialogo, rifiuta con cocciuta e inquietante determinazione ogni ipotesi di miglioramento del testo in discussione, rendendo drammaticamente trasparenti le vere ragioni del suo procedere. *(Commenti dal Gruppo PdL).* Vi è uno scenario che si intravede, alla fine di questo percorso. Questo scenario è né più né meno

Contro il procuratore di Caltanissetta Sergio Lari, il suo aggiunto Domenico Gozzo, il procuratore aggiunto di Palermo Antonio Ingroia, il sostituto procuratore di Palermo Gaetano Paci dal Gruppo PdL)* era pronto un attentato stragista di Cosa nostra, che le forze dell'ordine hanno fermato in tempo. A questi magistrati, a questi servitori dello Stato deve andare la solidarietà di tutto il Parlamento, ma la vera solidarietà è quella di farli lavorare in pace, con il tempo necessario, per assicurare alla giustizia i criminali di Cosa nostra. MONTI *(LNP).* Tempo! GARRAFFA *(PD)*. Con questo provvedimento non state aiutando la magistratura. In un momento in cui deve vincere il rispetto nella politica e nella magistratura...

così. Nel giorno in cui la Corte europea dei diritti dell'uomo dichiara inammissibile il ricorso di un Ministro del I Governo Berlusconi, condannato con sentenza definitiva per corruzione aggravata, così riconoscendo l'equità del giudizio cui egli è stato sottoposto, la maggioranza si accinge ad un ulteriore, devastante passaggio del suo cinico progetto di disarticolazione della giustizia italiana. Mentre questa maggioranza - tristemente ridotta al rango di mera esecutrice di ordini - parla di dialogo, rifiuta con cocciuta e inquietante determinazione ogni ipotesi di miglioramento del testo in discussione, rendendo drammaticamente trasparenti le vere ragioni del suo procedere.

Propongo due considerazioni ai colleghi della minoranza. Primo. Cosa avrebbero detto e dichiarato se la Corte europea dei diritti dell'uomo avesse ritenuto ammissibile quel ricorso, dopo quindici anni dai fatti? Secondo. Poiché credo in una sana alternanza, radice della democrazia, la domanda da porsi è: come mai, dopo quindici anni da quei fatti, al di là della responsabilità dei singoli, il Governo Berlusconi e il centrodestra hanno avuto e continuano ad avere il più largo consenso popolare nelle ultime elezioni (sopra il 60 Sarebbe meglio, più fisiologico (anche negli interessi dell'opposizione), meditare su questa domanda e fare un'opposizione

cortesia, colleghi. In quest'Aula, in un minuto di dichiarazione di voto, ogni senatore è libero di esprimere le proprie opinioni. Prego, senatrice esecutrice di ordini, mira a gridare al Paese che alla fine di questo percorso esiste un solo scenario: lo scempio della giustizia italiana. Di questo scempio vi assumete davanti al Paese tutta la responsabilità politica e morale. *(Applausi dal

una dichiarazione di voto Signora Presidente, mi associo ai colleghi con una breve dichiarazione. La ripetizione dei nostri interventi, letti di fronte ad una maggioranza tristemente ridotta a mera esecutrice di ordini, mira a gridare al Paese che alla fine di questo percorso esiste un solo scenario: lo scempio della giustizia italiana. Di questo scempio vi assumete davanti al Paese tutta la responsabilità politica e morale.

**Il Senato non approva.** per confermare quanto già sostenuto dai colleghi, ancorché purtroppo nel dileggio o peggio ancora nell'indifferenza. Noi siamo convinti di essere di fronte ad un cinico progetto che di fatto lede le libertà democratiche. A dispetto di ciò che accade, si parla di Governo dell'amore, di apertura e di disponibilità; intanto questa maggioranza, tristemente ridotta a rango di mera esecutrice di ordini, rifiuta con cocciuta e inquietante determinazione ogni ipotesi di miglioramento del testo in discussione, rendendo drammaticamente trasparenti le vere ragioni del suo procedere. Siamo di fronte ad uno scempio e di questo scempio questa maggioranza e l'intero Governo Berlusconi dovrà assumersi la responsabilità di fronte a tutto il Paese.

è evidente al Paese lo scempio che state facendo con questa legge. Vi assumete una responsabilità politica grandissima e lo state facendo proprio nel giorno importante in cui la Corte europea dei diritti dell'uomo dichiara inammissibile il ricorso di un Ministro del I Governo Berlusconi, condannato con sentenza definitiva per corruzione aggravata, riconoscendo così l'equità del giudizio cui egli è stato sottoposto. La maggioranza si accinge ad un ulteriore e devastante passaggio del suo cinico progetto che è quello di devastare il sistema della giustizia italiana. *(Commenti dal Gruppo PdL)*. Di questo vi assumete la responsabilità.

perché la sua domanda è degna di una risposta precisa: cosa avremmo fatto? Avremmo rispettato la decisione di un organo giudiziario, perché siamo avvezzi a rispettarne le decisioni, e avremmo continuato a sdegnarci per le lungaggini processuali proponendo, come stiamo facendo, rimedi idonei e non una legge come questa, che devasterà la giustizia italiana.

l'articolo 4 concerne la clausola di monitoraggio. Noi dall'inizio della discussione di questo disegno di legge segnaliamo la presenza tuttora di profili di illegittimità costituzionale. In particolare, avevamo segnalato che questo disegno di legge è assolutamente privo di copertura, e questo è in violazione dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. Infatti, il disegno di legge prevede all'articolo 1

comportano assolutamente necessità di ordine finanziario. Con il senatore Legnini avevamo presentato degli emendamenti proprio per provvedere alla copertura finanziaria; ci è stato risposto in maniera negativa sia in Commissione che all'interno di quest'Aula. Per contro, questo articolo 4, inserito successivamente dal Governo e dalla maggioranza, ci dà peraltro contezza del fatto che questa esigenza finanziaria era stata considerata positivamente dal Governo, tant'è vero che si incarica il Ministro dell'economia e delle finanze di assumere tempestivamente iniziative legislative per assicurare il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione. Ora, oltre alla irritualità istituzionale di una delega di questo tipo al Ministro dell'economia e delle finanze, rileviamo che nella sostanza ciò conferma i nostri dubbi di palese incostituzionalità.

assume le conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione». Sinceramente, non comprendo quale sia, non solo dal punto di vista squisitamente letterale,

sul bilancio del Ministero di giustizia di tutte le domande di equa riparazione che verranno presentate a seguito dell'entrata in vigore di queste disposizioni, che si applicano anche ai processi in corso.

per gli oltre 2.500.000 giudizi civili pendenti che hanno già superato la soglia della durata ragionevole del processo

Pinto, e quante unità di personale ci vorranno solo per le cancellerie presso le corti d'appello, per reggere il carico di lavoro determinato da questa norma, che fa diventare irragionevole - mi scusi il bisticcio di parole - la ragionevole

il disprezzo e persino i sorrisi ironici con i quali la maggioranza risponde ai nostri appelli e alle nostre dichiarazioni non nasconderanno la gravità di ciò che sta succedendo, l'esecuzione di un ordine scellerato: approvare una legge che mira a realizzare un solo scenario, la morte, lo scempio della giustizia italiana. Di questo noi non ci assumiamo alcuna responsabilità;, quelle politiche e quelle morali ve le assumete appieno

Signor Presidente, la ripetizione dei nostri interventi, pronunciati di fronte ad una maggioranza tristemente ridotta a mera esecutrice di ordini... ...*mira a gridare al Paese che alla fine di questo percorso esiste uno scenario solo: lo scempio della giustizia italiana. Di questo scempio vi assumete davanti al Paese tutta la responsabilità, sia politica che morale.

ordini. Quando noi diciamo che il Parlamento è paralizzato, non lo facciamo perché noi siamo opposizione e voi maggioranza. Voi dovete ritirare i vostri emendamenti e, peggio ancora, non potete votare quelli che presentate, cari colleghi. Ricordatevi di questo. È per questo che dello scempio che oggi state compiendo vi assumete la responsabilità davanti al Paese.

Presidente, colleghi, vi sono giorni in cui niente è più chiaro di una dichiarazione di voto universale. il giorno in cui la Corte europea dei diritti dell'uomo dichiara inammissibile il ricorso di un Ministro del I Governo Berlusconi, condannato con sentenza definitiva per corruzione aggravata, così riconoscendo l'equità del giudizio cui egli è stato sottoposto, la maggioranza si accinge ad un ulteriore, devastante passaggio del suo cinico progetto di disarticolazione della giustizia italiana. Vi è uno scenario che si intravede alla fine di questo percorso. Questo scenario è né più né meno che lo scempio della giustizia italiana. Lasciatemelo ripetere: lo scempio della giustizia italiana. Di questo scempio vi assumete davanti al Paese

è in essa. Nel giorno in cui la Corte europea dei diritti dell'uomo dichiara inammissibile il ricorso di un Ministro del I Governo Berlusconi, condannato con sentenza definitiva per corruzione aggravata, così riconoscendo l'equità del giudizio cui egli è stato sottoposto, la maggioranza si accinge ad un ulteriore, devastante passaggio del suo cinico progetto di disarticolazione della giustizia italiana.

parla di dialogo, rifiuta con cocciuta e inquietante determinazione ogni ipotesi di miglioramento del testo in discussione, rendendo drammaticamente discussione, rendendo drammaticamente trasparenti le vere ragioni del suo procedere. Vi è uno scenario che si intravede, alla fine di questo percorso.

dichiara inammissibile il ricorso di un Ministro del I Governo Berlusconi, condannato con sentenza definitiva per corruzione aggravata, così riconoscendo l'equità del giudizio cui egli è stato sottoposto, la maggioranza si accinge ad un ulteriore, devastante passaggio del suo cinico progetto di disarticolazione della giustizia italiana. Al dispiegarsi di tale cinico progetto assiste un pubblico esterrefatto e sgomento di avvocati, di personale giudiziario, di magistrati,

è sorto un problema tecnico. Da quando lei si è insediato in Presidenza, sentiamo una voce a 78 giri. Invito i tecnici a rimettere la puntina a 45 giri.

discutiamo introduce anche il tema delle giurisdizioni amministrative e contabili. Come ho già avuto modo di dire nel corso della precedente seduta, si è ritenuto che sia la pretesa punitiva dello Stato che la pretesa risarcitoria debbano essere contenute in termini circoscritti, pena la sanzione processuale. Pertanto, confermo l'emendamento, che varrà naturalmente per i processi futuri, in quanto la modifica entrerà in vigore dopo che questo disegno di legge

La ripetizione dei nostri interventi letti di fronte a voi, ad una maggioranza tristemente ridotta a mera esecutrice di ordini, mira a gridare al Paese che alla fine di questo percorso esiste un solo scenario: lo scempio della giustizia italiana. Di questo scempio vi assumete davanti al Paese tutta la responsabilità politica e morale. *(Applausi dal Gruppo* Signor Presidente, sinceramente non comprendo la ragione per la quale la maggioranza ha voluto introdurre questa norma che distrugge totalmente il giudizio davanti alla Corte dei conti degli amministratori e dei funzionari che si macchino di un reato molto più grave da un certo punto di vista - ad esempio, dalla prospettiva del federalismo fiscale - cioè quello di aver arrecato un danno alla finanza pubblica, alle finanze dello Stato, delle Regioni, dei Comuni, delle Province e così via. Non ne capisco sinceramente la ragione, perché peraltro questa disposizione - poi della norma transitoria, quando sarà oggetto di discussione, parleremo - distrugge distrugge il giudizio contabile e, quindi, rende di fatto impossibile la celebrazione dei giudizi di responsabilità degli amministratori il giorno in cui voi, con le vostre deleghe sul federalismo fiscale, trasferirete più competenze, più poteri di spesa agli enti locali. Quindi, è illogico, da un lato, devolvere al sistema delle autonomie maggiori competenze e un maggiore potere di imposizione fiscale e, dall'altro, non rafforzare i poteri di controllo della giurisdizione della Corte dei conti per verificare se quelle tasse, se quelle imposte, se quel prelievo fiscale che gli amministratori locali richiedono siano funzionali all'interesse pubblico oppure allo sperpero di risorse dei contribuenti. Questa è la cosa che non si capisce di ciò che state facendo, o meglio non la si capisce nella logica della coerenza di un progetto politico che dite di voler portare avanti con il federalismo fiscale. Si spiega in una logica diversa, che è tutta contingente: quella cioè di evitare che si possa celebrare in una determinata fase storica una serie di processi contabili. Ebbene, in questa logica quello che state facendo è assolutamente coerente. Disprezzabile politicamente, ma coerente. Da questo punto di vista, però, mi permetto di segnalare un paio di questioni, perché state varando una norma che è assolutamente fuori da qualsiasi criterio di costituzionalità. Infatti, non potete distinguere la durata di un processo davanti alla Corte dei conti a seconda della quantificazione del danno: questo è un espediente che serve solo ad accorciare alcuni processi e solo per l'applicazione della norma transitoria.

durano da più di due anni e che, siccome forse riguardano qualcuno che vi interessa, non avete alcun interesse a che vengano celebrati. Diventa più chiaro ciò che si sta facendo e verosimilmente può darsi che si individui una soluzione migliore rispetto a quella di distruggere l'intero sistema del giudizio della Corte dei conti. Perché voi, per fare questa porcheria, state sostanzialmente affidando al pubblico ministero presso la Corte dei conti poteri enormi. poteri enormi. Ma le leggete le cose che scrivete? State dicendo che la fase delle contestazioni che il pubblico ministero fa all'amministratore non rientra nel computo del periodo relativo alla prescrizione del processo: la tagliola scatta nel momento in cui l'atto di citazione in giudizio viene depositato presso la segreteria della sezione giurisdizionale della Corte dei conti, ma la fase precedente in cui il pubblico ministero raccoglie le prove sulla responsabilità contabile, attiva la Guardia di finanza (come è giusto che venga fatto), dispone di tutti i mezzi istruttori unilateralmente e poi chiede le controdeduzioni alla parte, ma senza alcun contraddittorio, questa fase è libera nel tempo, ha una durata verosimilmente illimitata e non è soggetta alla tagliola. Perché fate questo? Perché è una fase che non vi interessa, perché verosimilmente non avete alcun caso concreto a cui doverla applicare. Guardando questa norma a regime, mi chiedo

vi è un'assoluta disparità di trattamento con ciò che avete fatto sul giudizio penale, in cui si può discutere dei limiti di tempo, ma si è giustamente stabilita una virata anche per i giudizi in Cassazione. Ricordo a me stesso che le decisioni che la Corte dei conti prende in sede di appello sono ricorribili per Cassazione, però il termine del giudizio per Cassazione relativo alle decisioni della Corte dei conti non rientra nella ragionevole durata del processo, il che mi sembra una castroneria. tralasciando questo aspetto, secondo voi è possibile che la durata del giudizio contabile la stabilisca il pubblico ministero? Perché la quantificazione del danno la contestazione del danno è quella fatta dal pubblico ministero. Vi sembra normale che sia il pubblico ministero a stabilire se quel giudizio dovrà durare due o giudizio dovrà durare due o tre anni? È evidente che farà in modo che tutti i giudizi durino tre anni e alzerà il livello della contestazione del danno patrimoniale. E questo non va a detrimento del diritto di difesa? Non va contro l'interesse del contraddittorio e della tutela dei convenuti nel giudizio contabile?

gli adempimenti istruttori nel corso del giudizio. Ritenete solo che debba essere tolto dal computo dei due o dei tre anni e tempo conseguente ai rinvii chiesti dalla parte convenuta, che è una cosa giusta.

diverse sezioni, per avere un'indicazione univoca sul principio o sulla interpretazione della norma da applicare, il tempo necessario a che le sezioni riunite decidano viene calcolato nell'ambito dei due o dei tre anni.

chiede e dispone un'ordinanza istruttoria per accertare essa stessa direttamente se i fatti che sono portati in giudizio costituiscono causa di responsabilità erariale, queste ordinanze e per l'acquisizione della prova da parte della Corte dei conti non viene calcolato nell'ambito della durata del processo. Lo stesso per quanto riguarda la remissione alla Corte costituzionale, e così via. Allora, in buona sostanza, per salvare qualcuno da qualche processo davanti alla Corte dei conti, state sostanzialmente il processo contabile e - nella migliore delle ipotesi - state togliendo alla difesa dei convenuti il diritto di spiegare le proprie ragioni nell'ambito del giudizio,

di dimostrare se quelle risorse, quelle spese o quegli atti sono conformi o no all'interesse generale. Di questo non vi interessa nulla. E che non interessi nulla a voi poco importa; mi meraviglia invece che la Lega, che del federalismo fiscale ha fatto la propria battaglia principale, abbia consentito di distruggere uno degli strumenti fondamentali perché esso possa trovare attuazione.

sapete meglio di me che, allo stato attuale, il giudizio di responsabilità contabile è uno dei migliori dal punto di vista dell'efficienza e dell'efficacia. È tendenzialmente un processo *per tabulas*, quindi abbastanza facile da gestire da parte delle procure

Se in un procedimento ci sono «n» persone imputate per il medesimo fatto dannoso, questo importo massimo di 300.000 euro, ovviamente, si riduce *pro quota* per le singole persone. Ciò significa

Grazie,

Signor Presidente, tralascio la Corte europea dei diritti dell'uomo e il riferimento al cinico progetto che abbiamo ripetuto abbastanza e che credo sia stato recepito dai colleghi della maggioranza. passaggio relativo alla maggioranza tristemente ridotta al rango di mera esecutrice di ordini. Badate colleghi, questa è un affermazione pesante, un'affermazione grave,

avete ben capito che questa è una legge che devasterà la giustizia italiana! Vi state però assumendo l'onere e la responsabilità davanti al Paese di votarla, quando ben sapete che per ridurre i tempi della giustizia ci sono

Signor Presidente, signore e signori del Senato, non ho ben compreso che cosa abbia fatto oggi la Corte europea dei diritti dell'uomo. Mi pare di capire che abbia preso una decisione che ha fatto felice una parte della minoranza, quella rappresentata dal Partito Democratico. Ma al tacere di questo, io ho qui sentito questa minoranza che si è esercitata in un'elegante *tantra* ripetitivo,

desidero contribuire con la seguente dichiarazione, di cui ovviamente mi assumo in pieno la responsabilità storica, morale, civile e politica.

Sapete quali siano stati sempre l'orientamento e l'atteggiamento di questa Presidenza: di consentire a qualunque Gruppo, anche a fronte dell'esaurimento dei tempi, l'intervento di un minuto per garantire la libertà d'espressione e il diritto di parola nel merito dei provvedimenti. inutile sottolineare come questo minuto di parola sinora sia stato utilizzato non tanto per manifestare perplessità o valutazioni nel merito del singolo emendamento, ma per svolgere un'attività semiostruzionistica (non voglio definirla ostruzionistica). quindi i colleghi, da questo momento in poi, a chiedermi la parola soltanto nel caso in cui debbano intervenire nel merito dell'emendamento: in quel caso questa Presidenza non si sottrarrà alla propria consuetudine di garantire il diritto di parola. Nel caso in cui, invece, dovesse essere ripetuta una dichiarazione di voto che nulla ha a che vedere con l'emendamento e che quindi va in discrasia con quello che è stato il mio orientamento, vi prego di evitarlo, perché il diritto di parola di un minuto lo garantisco sempre, ma purché vi sia un intervento nel merito del provvedimento, anche perché siamo alla fine.

A voler analizzare il senso della sua dichiarazione d'intenti (non so se è un provvedimento o altro), si introduce, secondo ciò che lei ci ha detto or ora, una facoltà, che non credo sia prevista dalla disciplina che regola le nostre attività, di intervento nel merito delle dichiarazioni di voto dei singoli parlamentari, che davvero, col dovuto rispetto, credo non rientri nelle sue prerogative.

la qualità dell'amministrazione della giustizia in Italia da oltre trent'anni e altrettanto fa da un quindicennio la Corte europea dei diritti dell'uomo. Quindi le responsabilità credo siano ampiamente condivise e, ahimé, mai ritenute

vista l'attenzione - quattro per la dichiarazione di voto sulla norma transitoria e, se lei lo ritiene possibile, cederò 10 minuti ai colleghi del Partito Democratico e dell'Italia dei Valori, per consentire di sviluppare le loro osservazioni sul merito delle questioni.

Da parte della Presidenza non vi è stata mai, né vi sarà mai, la volontà di strozzare il dibattito o la libertà di parola dei colleghi, purché - vivaddio - si entri nel merito dell'emendamento che si discute, non del provvedimento in senso lato.

sui 72 previsti. Con il processo breve quanti mafiosi verranno liberati? Un collegamento audiovisivo, un trasferimento saltato: si darebbe quindi la stura a quella che io e molti altri chiamiamo la mega-amnistia. Colleghi della maggioranza, vergognatevi!

Presidente, onorevoli colleghi, vorrei riprendere un invito rivolto alla maggioranza e al Governo nella conclusione del dibattito generale. Abbiate il coraggio di votarvi senza una patetica ipocrisia una norma costituzionale a maggioranza, che è ampia, come l'avete in quest'Aula

Signor Presidente, farò una breve dichiarazione di voto. La ripetizione dei nostri interventi, letti di fronte a una maggioranza tristemente - soprattutto per la vostra dignità ridotta a mera esecutrice di ordini, mira a gridare al Paese che alla fine di questo percorso esiste un solo scenario: lo scempio della giustizia italiana. Di tale scempio vi assumete oggi, davanti al Paese, tutta la responsabilità politica e morale.

non ripeterò le parole che hanno detto i miei colleghi, ma una cosa ci tengo a dirvela. Io mi auguro che questa responsabilità grossa che vi prendete nei confronti del Paese non voglia significare niente per quanto riguarda le morti sul lavoro e il disastro ferroviario di Viareggio. Come ho avuto occasione di dire al senatore Valentino in Commissione, mi auguro che non ci siano ripercussioni in tal senso, perché allora la responsabilità sarebbe elevata all'ennesima potenza. Signor Presidente, ho parlato della Sicilia, adesso parliamo dell'Europa.

Al dispiegarsi di questo cinico progetto assiste un pubblico esterrefatto e sgomento di avvocati, di personale giudiziario, di magistrati, di professionisti della sicurezza e, soprattutto, di cittadini. Mentre questa maggioranza - tristemente ridotta al rango di mera esecutrice di ordini - parla di dialogo, rifiuta con cocciuta e inquietante determinazione ogni ipotesi di miglioramento del testo in discussione, rendendo drammaticamente trasparenti le vere ragioni del suo procedere. Vi è uno scenario che si intravede, alla fine di questo percorso. Questo scenario è né più né meno che lo scempio della giustizia italiana. Lasciatemelo ripetere: lo scempio della giustizia italiana. Di questo scempio vi assumete davanti al Paese tutta la responsabilità, politica e morale. Vergognatevi di nuovo!

a prescindere dal fatto che non stiamo facendo interventi ostruzionistici, ma semmai di protesta politica perché la maggioranza non si esprime nel merito dei nostri emendamenti. E questa è una cosa diversa. Abbiamo appena respinto - mi dispiace di non essere riuscita ad attirare l'attenzione dei colleghi

milioni. La maggioranza non deve offendersi se diciamo che siete ridotti ad essere esecutori di ordini o di dimostrazioni di prove d'amore che vi ha chiesto il presidente Berlusconi. Questo emendamento non c'entrava niente con tutto il resto:

Presidente, colleghi, avremmo voluto stupirvi con effetti speciali, ma l'impegno della nostra lotta di liberazione per la maggioranza non conosce soste. Mi permetta solo di dirvi: no al processo breve, no alle briglie corte, libertà per i detenuti politici, liberateli senza condizioni!

nelle nostre dichiarazioni che siamo di fronte ad uno scempio grave della giustizia italiana. È necessario gridare al Paese che questo percorso va cambiato e che vi è una maggioranza che si assume la responsabilità

c'è il merito per dire che stiamo commettendo un grave errore che non semplifica la nostra giustizia. Credo che vada ribadito: viene fatto scempio della giustizia italiana.

Presidente, colleghi della maggioranza, voi manifestate fastidio per il fatto che reiteriamo i nostri interventi, ma il fatto che cerchiamo di concentrarci sulla circostanza che oggi è il giorno in cui la Corte europea dei diritti dell'uomo dichiara inammissibile il ricorso di un Ministro del I Governo Berlusconi, condannato con sentenza definitiva per corruzione aggravata, non è estraneo allo scempio che state compiendo parlando fuori di qui di dialogo ed essendo in realtà in questa sede soltanto meri esecutori di ordini che arrivano dall'alto. Come diceva prima giustamente la senatrice Adamo, anche quando ci sono emendamenti di buon senso li rifiutate. Il problema è che state facendo uno scempio; dovete averne la responsabilità e la consapevolezza, e noi non ci stancheremo, con l'unica maniera che abbiamo a disposizione, di ripeterlo e di ribadirlo fino alla fine.

Grazie

perché vogliamo gridare al Paese che, alla fine di questo percorso che voi ostinatamente volete perseguire, esiste un solo scenario: lo scempio della giustizia italiana.

e all'Unione europea, che riconosce l'universalità dei diritti e l'equità del giudizio a livello europeo. Di fronte a ciò

Presidente, intervengo per un richiamo al Regolamento su una questione che ritengo essere di un qualche rilievo; quindi, la prego

e affronta la materia del regime transitorio del cosiddetto processo breve. Questa norma che la maggioranza ha votato poco fa ci dice che le norme sul processo breve si applicano, per i processi pendenti, a quelli relativi alla cosiddetta responsabilità penale dell'impresa e delle persone giuridiche. Questo il testo che abbiamo votato mezz'ora fa.

che presentano evidenti profili di preclusione. È questo il punto del richiamo al Regolamento, in particolare all'articolo 97,

dall'Aula un emendamento riguardante la tutela penale dei diritti di proprietà industriale (la contraffazione, l'alterazione e così via). Poiché erano stati presentati due emendamenti che affrontavano il medesimo argomento, uno dal relatore

attenzione: quindi le chiedo di dichiarare formalmente preclusi gli emendamenti 4.0.1001 e 4.0.1001/300.

è il tentativo di introdurre un ulteriore articolo 4-*bis*. Io non penso che questi errori accadano per caso. Io ritengo che la buona coscienza dei colleghi

a chi questa norma chiedeva, ma che nella sostanza abbiano voluto proporre qualcosa che non è più proponibile, se non sovvertendo il nostro Regolamento. Rispettiamo il Senato!

Credo che l'intervento sia suggestivo, ma sostanzialmente irrilevante. che la questione non sia obiettivamente strumentale. Qui c'è un problema di garanzia e di forma del procedimento legislativo, di ciò che si esamina, di ciò che si vota, e la numerazione e la la classificazione delle norme in articoli è funzionale a far sì che il parlamentare, nel momento in cui si esprime, abbia consapevolezza della consequenzialità logica di ciò che si approva, di ciò che viene soppresso e di ciò che viene approvato.

in Aula dal relatore. La riscrittura di questa disposizione, infatti, è stata fatta in Aula dal relatore successivamente alla classificazione come articolo 4‑*bis* della norma di cui parlava il collega Legnini. problema non è quello di dare un'interpretazione autentica: è evidente che questa è un'altra disposizione e che tutto questo non può che comportare le conseguenze che sul piano regolamentare il collega Legnini ha esposto. Siamo infatti in presenza di due disposizioni, di cui una successiva all'altra, che presentano la medesima numerazione. E tutto ciò non è frutto di un refuso, ma di una chiara intenzione, verosimilmente, di intervenire successivamente con una norma che sostituisce la precedente o che comunque è in concorrenza essa. Siamo cioè in presenza di due articoli 4‑*bis*, il che non è irrilevante dal punto di vista della garanzia del Parlamento e dei singoli parlamentari nell'esercizio del loro diritto-dovere di voto delle singole proposte. Signor Presidente, non ho uno lunga esperienza parlamentare, però, per quanto ho visto sia alla Camera che al Senato, ogni volta che si aggiungono nuovi articoli la numerazione è sempre la stessa. (ad esempio, 4-bis). Si tratta di valutare piuttosto se si tratta di materie diverse o della stessa materia.

che "le previsioni del comma 1 si applicano anche alle ipotesi di responsabilità amministrativa degli enti di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231".

è una giornata particolarmente disagevole per noi che ci occupiamo di diritto. L'unico momento di sollievo è nel fatto che con questo emendamento la maggioranza si è assicurata un ottimo giudizio di incostituzionalità. A pagina 117 abbiamo poc'anzi approvato l'emendamento 1.1001, che disciplina

Si tratta di norme processuali e giustamente voi, che ben conoscete l'articolo 11 delle preleggi che

per ricorrere all'indennizzo, ai sensi della legge Pinto, avete previsto il rispetto del principio del *tempus regit actum*, perché avete scritto: «Alle domande di equa riparazione proposte anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge

Ma nello stesso provvedimento - ecco il criterio di profonda irragionevolezza che vi farà naufragare nella incostituzionalità - inserite un'altra norma processuale con cui ritenete di poter applicare con effetto retroattivo la tempistica di un processo sviluppatosi nel passato, quando non esisteva detta tempistica.

Il giudice della Cassazione, processo in corso, dovrà verificare se siano decorsi più di due anni dal provvedimento con cui il pubblico ministero ha esercitato l'azione penale senza che sia stato definito il giudizio. Facendo questa verifica, qualora

prevedete che nel giudizio di Cassazione, attraverso la norma transitoria, il giudice della Cassazione vada a verificare quanto è successo in primo grado, cioè quello che è successo alcuni anni fa, e accerti ora per allora se la durata di quel processo già fatto abbia rispettato i termini oggi introdotti. Questa è una norma palesemente incostituzionale. Chiedo poi al relatore di capire. Si è fatto un riferimento temporale alla data di entrata in vigore dell'indulto. Questo Questo riferimento temporale, però, era stato già utilizzato nella legge n. 125 del 2008, quella "blocca processi", ma con quale portata? In quella legge approvata da questo Parlamento venivano differenziati i processi sulla base della legge che aveva introdotto l'indulto, tenendo conto però della pena eventualmente da infliggere che può essere contenuta nei limiti di cui all'articolo 1. In sostanza, era un riferimento: si sospendono i processi la cui pena si prevede che rientri nei tre anni previsti dall'indulto. Questa è la legge che abbiamo approvato, la n. 125 del 2008. Il relatore inserisce lo stesso discrimine temporale,

meno un giorno. Quindi, il discrimine del prima e del dopo non ha una ricaduta giuridica come l'aveva nella legge n. 125 del 2008. È solo un riferimento temporale che non riguarda i processi

Ma non vi rendete conto dell'enorme disparità di trattamento tra il cittadino che commette un reato prima del 2 maggio 2006, ma che non ha avuto il processo, che nasce dopo, perché dopo partono le indagini, e viene imputato, per cui in questo caso godrebbe del processo di durata massima di due anni e il cittadino che, invece, commette un reato

dal nostro punto di vista l'approvazione da parte della maggioranza di questa norma transitoria è dirimente per il voto contrario a questo testo. infatti, che siamo in presenza di una norma che, rispetto al vecchio testo della disposizione transitoria, riduce il numero dei processi in corso cui si applicano le disposizioni e individua in maniera "chirurgica" una serie di processi che si estinguono nonostante le norme processuali nuove debbano valere per il futuro.

mi riferisco ai colleghi della Lega e ai tutori della certezza della pena presenti all'interno del Popolo della Libertà, che nella scorsa legislatura, giustamente - dal loro punto di vista - hanno gridato allo scandalo per l'approvazione del mini-indulto. Intendo spiegare loro che quello che stanno votando oggi è non solo un indulto, ma una vera e propria amnistia per una serie di reati. Procediamo per ordine.

che riguardano i reati commessi fino al 2 maggio 2006 - data stabilita per l'applicazione dell'indulto se hanno superato il limite biennale si estinguono per prescrizione. E poiché a questa regola si applica anche il principio del *ne bis in idem*, quindi c'è una preclusione, per per gli stessi fatti, con riferimento alle stesse persone, ad agire con un altro processo, siamo in presenza non di una prescrizione processuale, ma di un condono tombale, di un'amnistia. Ora, è assolutamente evidente la disparità di trattamento di cui ha parlato il collega Li Gotti, che quindi consacra la violazione dei principi fondamentali della nostra Carta costituzionale; come è altresì evidente che tutto questo determina la violazione ancor più marcata di quelle disposizioni costituzionali che garantiscono il diritto di difesa. Ciò è evidente per tutte quelle parti civili, quelle vittime di reato

qui state votando una roba che è quattro volte l'indulto. Anche qui, diamo alle cose un nome e un cognome, perché poi, non vi sarà consentito di fare gli sbruffoni con la certezza della pena. Ma quale certezza della pena? Di quale certezza della pena state parlando?

le argomentazioni portate mi convincono, ma fino ad un certo punto. Poiché quella disposizione che reca la stessa numerazione di questa che stiamo votando è stata già approvata in precedenza e poiché in sede di quel voto non si è precisato che si trattava di un'integrazione (quella di cui stiamo parlando ora), è chiaro che l'Aula ha votato un testo e che l'emendamento 4.0.1001 dovrebbe formalmente e sostanzialmente restare precluso. Questa poteva essere un'ipotesi per evitarvi l'umiliazione di fare un condono tombale ed un'amnistia, che è qualcosa di più, molto più grave e meno trasparente ed onesto nei confronti dei vostri elettori,

E potete continuare a mugolare, perché tanto, fino a quando ho tempo, parlo e non mi faccio turbare dai vostri mugolii e dai vostri mal di pancia. *(Applausi perché avete fatto il condono tombale per i vostri amministratori che sperperano il denaro pubblico, salvo poi dire agli elettori che farete il federalismo fiscale, per cui i cittadini avranno un maggior controllo. Ma che tipo di tutela ha il cittadino, quando, se il sindaco o l'assessore sprecano il denaro pubblico, non si può andare alla Corte dei conti? E oggi fate finta di niente e vi girate dall'altra parte, rispetto ad un'amnistia che state votando per reati commessi prima del 2 maggio 2006, nei confronti dei quali, quando nella passata legislatura si votò l'indulto, avete sfoderato i vecchi cappi e li avete portati in giro per il Paese: vi dovete solo vergognare! Signor Presidente, siamo giunti al vero motivo di tutto questo disegno di legge e, per così dire, al cuore del provvedimento, perché per il Governo e per la maggioranza era ed è necessario salvare il Presidente del Consiglio dei ministri dai suoi processi penali.

vi siete allargati e avete provato a salvare anche un vostro Ministro e un vostro sindaco da ben cinque processi contabili. Ecco allora che, alla norma transitoria a favore del Presidente del Consiglio dei ministri, anche in materia di processo contabile aggiungete una norma che vale a salvare alcune altre vostre persone, come indicato.

se fossero la stessa cosa e non rendendovi conto dei guasti che andate a creare anche all'interno del processo contabile, come abbiamo ricordato poco fa. Per quanto riguarda il processo davanti alla Corte dei conti, dei conti, di fronte alla norma che avevate introdotto in prima battuta, si era ravvisata la necessità di prevedere un regime transitorio che rendesse inapplicabili le nuove disposizioni a processi in corso in primo o in secondo grado al momento di entrata in vigore della legge. perché, in assenza di questo regime transitorio, per numerosi processi pendenti sia in primo grado che in appello si verificherebbe - come abbiamo già detto - l'effetto estintivo dell'intero giudizio, non del singolo grado, con rilevanti perdite per l'erario, come effetto immediato dell'entrata in vigore della legge e senza spazio alcuno per possibili accelerazioni dei dibattimenti. Con la norma transitoria in materia di processo contabile, ricordo anche che sono in contestazione per due illustri personaggi della maggioranza - un Ministro e un sindaco - circa 500 milioni di euro.

dunque ove sia stata esercitata l'azione penale - per reati per così dire indultabili, puniti con pene inferiori ai dieci anni, qualora siano decorsi più di due anni dall'atto dell'esercizio penale senza la conclusione del primo grado di giudizio. Qui c'è un'evidente discrasia del termine di prescrizione, perché ordinariamente si parla di tre anni a regime, ma in questo caso, per una determinata categoria di reati,

e, come abbiamo detto anche durante la discussione generale, è a favore della persona del Presidente del Consiglio dei ministri. Vi chiediamo dunque di avere il coraggio di dirlo e di dichiararlo, perché in prima battuta avete rimediato ad alcuni guasti pesanti, anche dal punto di vista della legittimità costituzionale: infatti intervenuti con una pulizia, seppur superficiale, e con l'eliminazione dei vizi costituzionali più evidenti, che a nostro parere non avrebbero consentito nemmeno la firma del Presidente della Repubblica.

Nello scrivere le norme sul regime transitorio, pur riducendo il numero dei processi sottoposti a questa normativa, non vi siete scordati del motivo vero per cui siete andati avanti e avete presentato il disegno di legge. Pur facendo entrare in vigore le norme sul cosiddetto giusto e breve processo solo dopo l'entrata in vigore della legge, i processi a carico del Presidente del Consiglio dei ministri vengono cancellati subito. Complimenti: operazione riuscita! Decidete di sfasciare il sistema processuale penale pur di cancellare i processi penali contro il Presidente del Consiglio; create dei danni all'interno del processo contabile pur di creare un vantaggio a un vostro Ministro e a un vostro sindaco. Complessivamente si è parlato di un'amnistia strisciante: io parlo di un'amnistia anche permanente. Complimenti a voi e al vostro senso dello Stato!

della limpidezza del procedimento stesso e della possibilità per ciascun parlamentare di esercitare compiutamente il proprio ufficio: deve essere governato cioè dalla regola che bisogna, in ogni momento, essere in grado di comprendere quale sarà l'esito finale di ciascuna votazione, sia che essa registri un voto maggioritario positivo dell'Aula, sia che si registri un voto negativo. Torno quindi sulla questione che è stata sollevata dal senatore Legnini me lo consenta, Presidente - trovo sia stata da lei liquidata con una certa approssimazione e forse con qualche disattenzione nei confronti delle ragioni opposte da questa parte politica.

che rechi una disciplina solo parziale del regime transitorio. L'obiezione che lei ha opposto al senatore Legnini

con il temperamento dovuto al fatto che siamo ancora nel corso del procedimento legislativo non può essere adoperato in ogni sua pienezza, secondo cui

e ciò preclude l'emendamento 4.0.1001, che ha l'identico oggetto, ancorché parziale, perché nulla esclude che si sia voluto, in sede di ripensamento, presentare un emendamento che abbia appunto un contenuto parziale piuttosto che quello più vasto, peraltro dell'emendamento successivo.

peraltro, mi permetto di aggiungere che nella grande confusione, ma anche nella grande spadroneggiante libertà che il relatore e il Governo si sono presi nell'esame di questo provvedimento potevano almeno prendersi il disturbo

ha avuto successo di pubblico perché allora, nel 1893, almeno banchieri e politici andavano in galera e cadevano i Governi,

approvata il 29 dicembre 2005, i processi vennero estinti e gli autori di quelle gravissime frodi ai danni di decine di migliaia di risparmiatori

(...)», voi tutelate i banchieri. Lo ha ricordato la senatrice Adamo: quei derivati avariati appioppati al Comune di Milano che si estingueranno. Noi

vi mostreranno eterna gratitudine, ma non lo faranno i risparmiatori truffati, ossia quel milione di famiglie che piangono lacrime e sangue perché i banchieri le hanno frodate.

Non entrerò nel merito del provvedimento, perché lo farà il presidente Gasparri domani. E non entrerò nel merito delle strategie dell'opposizione, che ha inscenato in Aula una protesta, ovviamente legittima. Ma mi permetterete di dirvi - e questo è un giudizio politico che non vuole in nessuno modo essere offensivo - che ai nostri occhi

ce lo dovrebbe insegnare. Tuttavia, in questo caso, Signor Presidente, sul provvedimento in esame è stato seguito un *iter* che ha coinvolto profondamente il Gruppo, che ha portato questo Gruppo a lavorare con serietà

è stato interprete in quest'Aula con le sue iniziative. Abbiamo dato una prova di maturità. In democrazia, signor Presidente, ci sono dei momenti nei quali la maturità si esprime anche rimanendo nei banchi e non accettando le provocazioni. Questo non significa accettare di essere qualificati come pecore

serrare le fila in difesa del vostro Governo e della vostra maggioranza, nel momento in cui noi compivamo un'opera di protesta seria; avete rivendicato con orgoglio la vostra iniziativa e la vostra resistenza. Mi permetta, signor Presidente, di essere oggi orgoglioso della nostra maggioranza e del nostro comportamento e di ringraziare il relatore, i membri della Commissione giustizia e tutti i senatori che hanno partecipato a questa giornata parlamentare.

Noi, senatore Quagliariello, abbiamo fatto, come potevamo, un lavoro parlamentare di denuncia; non avevamo la possibilità di fare altro. Noi abbiamo semplicemente e soltanto denunciato - lo facciamo anche in questo momento e permetta di farlo

piangeranno molti italiani. Piangeranno le vittime, piangeranno i cittadini che aspettano il risarcimento del danno, per procedimenti che verranno interrotti a causa di una legge che ha un obiettivo diverso da quello che avete sbandierato in questa settimana di lavori. Mi permetta ora di dirle, signor Presidente, qualcosa che invece riguarda il modo con cui lei ha presieduto l'Assemblea durante i lavori relativi a questo disegno di legge. Lei ha avuto, nei confronti dell'opposizione, un atteggiamento che io non condivido e non approvo. Lei ha avuto nei confronti dell'opposizione un atteggiamento negativo, davanti a nostre richieste legittime. Le ho già detto, signor Presidente, e mi permetta di ripeterglielo...

Molta prudenza anche in relazione all'oggetto di questo provvedimento, che richiamava la Presidenza del Senato, eletta da una maggioranza che presenta il provvedimento con obiettivi specifici. Noi sappiamo quali sono i motivi per i quali il provvedimento è stato presentato ed è stato da voi votato. Signor Presidente, io penso - mi permetta di ripeterglielo - tener conto anche di questo nella conduzione dei lavori dell'Aula. Lei ha interpretato il Regolamento varie volte. Ma mi permetta di dirle, molto sinceramente e molto francamente, che lei ha interpretato il regolamento secondo la regola: «quello che io decido deve funzionare per l'Aula». Lei non ci ha convinto. Non ci ha convinto quando ha cercato di spiegare per quale motivo una Commissione è stata incaricata di esaminare un testo senza potersi esprimere su quel testo. Non ci ha convinto poco fa, signor Presidente, quando ha dichiarato - poi fortunatamente si è corretto nel comportamento - che noi avremmo dovuto

se noi avessimo detto qualcosa che non corrispondeva a quella regola. Adesso ha dichiarato ammissibile un emendamento che era chiaramente inammissibile, per ragioni che non ripeto e che molto bene hanno esposto i senatori Legnini e D'Alia e la senatrice Finocchiaro.

ai processi in corso di primo grado, salvo qualche eccezione che riguarda i giudizi d'appello, così come sono stati definiti in precedenza. Non voglio polemizzare con il collega Quagliariello, ma pacatamente vorrei ricordare che il nostro Gruppo parlamentare ha tenuto anche nel merito un atteggiamento diverso; lo ha fatto perché riteniamo che se non vi fossero state queste due disposizioni transitorie e finali, che ovviamente sono funzionali all'esigenza di sterilizzare il conflitto che oggi c'è tra Presidente del Consiglio e la magistratura, questo testo dal nostro punto di vista sarebbe sarebbe stato votabile, e non perché non riconosciamo la fondatezza almeno in parte dalle argomentazioni che il Presidente del Consiglio ha prodotto, ma perché riteniamo che se lo si vuole realmente - cominciamo ad avere il dubbio che nella vostra metà campo non lo si voglia realmente

Almeno seguiamo le regole che la Costituzione ci dà per affrontare questo tema. Possono essere modeste rispetto alle esigenze generali della coalizione che, visto che ci si trova, ritiene che siano tutti Berlusconi, quando non è così, per quanto ci riguarda se voi aveste voluto affrontare questo tema noi avremmo concorso a farlo. Siamo fiduciosi del fatto che ciò possa avvenire in seconda lettura alla Camera se ripulirete il testo di tutte quelle questioni che con la ragionevole durata del processo non hanno niente a che vedere. tutte quelle questioni che non servono e non sono funzionali ad attribuire pienezza di diritto al cittadino nel vedersi giudicato in tempi certi e con tutte le garanzie di difesa. Quello che sta avvenendo qui - purtroppo, dico io - in parte comprende le cose che ha detto lei e che condivido, ma in gran parte comprende una serie di materie estranee che, sotto le mentite spoglie di una mirabile regia tecnica e processuale, utilizzano questo tema per affrontare altre questioni, che si ha la voglia di trattare, ma in altra sede, e in maniera forse più efficace e più comprensibile da parte di quella maggioranza degli elettori che vi vota e vi ha dato il mandato di governare. Siccome si parla tanto della cosiddetta politica dei due forni, dico che la vera politica dei due forni è quella di chi dice una cosa all'elettore, ne prende il voto, e poi nelle Aule parlamentari ne fa un'altra. Su questo vi inviterei ad una riflessione più serena e pacata che, purtroppo, qui in Senato, non è stato possibile fare nonostante chiudiamo questo provvedimento complesso stasera alle ore 19, pur avendo in Conferenza dei Capigruppo fissato a domani alle ore 12 il termine per il voto finale. Non si può neanche contestare alle opposizioni di aver ostacolato, rispetto ai tempi concordati dei Capigruppo, l'esame del provvedimento. Semmai siamo noi a poter esprimere una doglianza: con questo gioco delle tre tavolette ci siamo ritrovati in Aula un testo totalmente diverso da quello che ci avete imposto con tempi rapidi di votare in Commissione, non consentendoci di approfondire tutta una serie di aspetti. Questo certamente ha strozzato il dibattito e l'approfondimento. Ma non vi è bastato: avete preteso non solo di cambiare il testo, ma anche di imporre il voto e la discussione solo su quelle due o tre questioni che il relatore con l'ultimo maxiemendamento, sbagliando la successione degli emendamenti, come ha detto la collega Finocchiaro, ha prodotto in quest'Aula. Queste sono le questioni che con grande serenità vi diciamo, che ci rammaricano, ma che non potranno che farci votare contro questo provvedimento così com'è: se lo cambierete alla Camera troverete il nostro sostegno. Presidente, domani il Ministro della giustizia verrà in quest'Aula e verosimilmente si eserciterà nel gioco delle tre carte. cioè a dire che questa giustizia non funziona e come vorrebbe migliorarla, mentre nelle ore antimeridiane voi andrete ad approvare questo sconcio logico, giuridico, etico, sociale e politico.

perché ci sia un momento di resipiscenza operosa per non licenziare un testo cattivo, che fa disonore all'intero Parlamento; un testo certamente incostituzionale - noi lo diciamo e lo gridiamo - che poi la Corte lo annullerà tra qualche mese e voi griderete, come al solito, al complotto, alle toghe rosse, alla giustizia politicizzata. Se scriveste norme un po' migliori e più corrette, e non soltanto per difendere il Presidente del Consiglio dai suoi problemi giudiziari, probabilmente riusciremmo a scrivere norme condivise insieme per il bene del Paese. Grazie, signor Presidente.

Avremmo più sicurezza per i cittadini o più insicurezza? Avremmo, Presidente, più razionalità o più disordine nel funzionamento della giustizia? Avremmo più parità dei cittadini

peggiorerebbe il contesto della giustizia. Non credo, Presidente, che sia stata allora una buona prova per il Senato concludere questi lavori trovandosi di fronte a due alternative: sperare che questo provvedimento venga insabbiato alla Camera mentre ne vanno avanti altri, oppure rassegnarsi alla circostanza che nel nostro Paese la

lo ha sottoscritto. E lo faremo perché dopo oltre dieci anni finalmente si inizia a dare attuazione ad una norma della nostra Costituzione, quella che voi spesso definite la Bibbia civile. La Costituzione ci chiede ci chiede una legge che assicuri la durata ragionevole dei processi; questa legge non c'era fino a oggi, domani colmeremo un vuoto presente in questo ordinamento da oltre dieci anni. Finalmente, daremo attuazione alla Carta costituzionale, che dal 1999 è rimasta inattuata sul punto. Sapete bene che questa riforma è maturata nei vostri ambienti dottrinari, è maturata dentro di voi. Abbiamo elencato tutti i progetti ed i disegni di legge utilizzati per redigere il disegno di legge Oggi siete costretti a rinnegare voi stessi! La sinistra è costretta a rinnegare se stessa, per non approvare una legge che va nell'interesse di tutti i cittadini. Voi non volete le leggi *ad personam*, volete le leggi *contra personam*. E questa legge non va contro una persona, ma va nell'interesse di tutti i cittadini!

viola un diritto dell'uomo. In quest'Aula, sentiamo spesso citare la Convenzione europea per i diritti dell'uomo per i Rom, per gli immigrati, ma non per i cittadini di questo Paese. Anche loro hanno una dignità umana che deve essere tutelata! *(Applausi dai

con il quale si chiede di sapere quali sono le motivazioni che ancora si frappongono all'accoglimento della richiesta di riconoscimento dello stato di crisi del comparto agroalimentare, avanzata dalle Regioni Basilicata, Sicilia, Sardegna, Abruzzo e Puglia, che appare oggi, allo stato degli atti, l'unica effettiva possibilità di vedere temperati gli effetti di una crisi inedita e senza precedenti. e per tali ragioni mi auguro

alla Presidenza del Consiglio dei ministri e ai Ministri competenti per gli adempimenti conseguenti.

L'interrogazione in questione chiede in particolare informazioni relativamente a tempi e costi per il rinnovo del permesso di soggiorno dei cittadini extracomunitari presenti

il 22 dicembre dello scorso anno. Credo sia quanto mai urgente avere dei chiarimenti relativamente, in particolare, ai tempi di rilascio del permesso di soggiorno, visto e considerato che oltre mezzo milione di cittadini non italiani presenti hanno un lavoro ma, in mancanza di detto permesso, non possono necessariamente godere dei diritti che, invece, il nostro ordinamento - e spero che la Lega sia con noi per chiederne il rispetto loro conferirebbe. Perché venga data una risposta oltre 300 extracomunitari, in particolare dell'Africa occidentale e dell'Asia, hanno avviato uno sciopero della fame a staffetta che è ancora in corso in queste ore. Spero che i Ministri competenti vogliano risolvere questo *rebus* in tempo utile perché poi si possa passare alla regolarizzazione di centinaia di migliaia di persone.